Abbiamo quindi un certo ingorgo nei nostri lavori di Commissione e avremmo bisogno, lo dico a nome di tutti i Gruppi della 5a,

(forse anche insieme alla 6a per quanto riguarda il decreto fiscale ma certamente per il decreto terremoto) di poter lavorare. La Commissione è già convocata oggi pomeriggio e lunedì.

Presidente, noi non abbiamo obiezioni di merito perché concordiamo sul principio e sul contenuto, avendo come priorità quella di dare soluzione ai problemi legati

nell'auspicio che l'Assemblea possa accettare la trattazione immediata del disegno di legge sul vino. Si tratta di un provvedimento, come credo i colleghi sappiano, da lungo tempo atteso da tutta la filiera, che ha anche lavorato molto intensamente prima con i colleghi della Camera dei deputati e, poi, anche con la nostra Commissione. La nostra Commissione si è già espressa all'unanimità su questo provvedimento. Voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno compreso da subito l'utilità di un lavoro accelerato che permettesse di approvare il provvedimento senza emendamenti, come era nostra intenzione. Tutte le forze politiche

un emendamento e ciò rende inevitabile una terza lettura dopo la nostra auspicata approvazione. Mi rendo conto che devo chiedere la comprensione dei colleghi della Commissione sanità che, a loro volta, avevano e hanno svolto un importante lavoro sul provvedimento di cui ieri abbiamo cominciato l'esame e di cui era prevista la continuazione questa mattina. l'Assemblea accettasse l'inversione dell'ordine del giorno, credo che potremmo procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge sul vino, tenuto conto che sono stati presentati pochissimi emendamenti e, quindi, la votazione potrebbe avvenire in tempi rapidi.

legato all'articolo 74, che ha portato a un certo cambiamento di rotta, grazie all'attenzione che il Senato ha

Presidente, noi abbiamo espresso il nostro consenso e siamo assolutamente convinti che si debba procedere così. Però, quanto ci ha detto il presidente Tonini questa mattina deve sollevare l'attenzione della Presidenza su un particolare. Come Commissioni

si avvia verso l'ennesimo voto di fiducia, signor Presidente, sarebbe stato bene evitare il passaggio nelle Commissioni, venire direttamente in Assemblea per il voto di fiducia e, alla prossima riforma, abolire definitivamente lo stesso Parlamento.

plastica dimostrazione dell'importanza del Senato e del bicameralismo, laddove con questo passaggio noi abbiamo la possibilità di correggere un errore,

noi stiamo dimostrando che così non è e che, probabilmente, si farebbe un errore se si proseguisse con questa riforma.

prendo atto con grande soddisfazione che l'Assemblea ha riconosciuto l'importanza di questo provvedimento, quindi deposito agli atti la mia relazione illustrativa sui vari articoli e mi limiterò a evidenziare le novità più significative

per la 9a Commissione, ma questa è particolarmente significativa. Ringrazio anche il vice ministro Olivero che ha seguito l'intero *iter* del provvedimento, rendendosi disponibile ad accogliere tutte le sollecitazioni provenienti dalla Commissione. Il disegno di legge ha avuto una lunga gestazione alla Camera, in un confronto complesso e articolato con tutte le rappresentanze del settore vitivinicolo e ciò ha rappresentato un successo per la condivisione ampia e convinta che abbiamo potuto constatare anche direttamente nelle audizioni e che ha convinto tutti a non ostacolare o rallentare il suo percorso. È un provvedimento concertato, capace di unire il mondo dell'economia con quello della politica e ritengo che questo sia un segnale che fa bene all'Italia. Passando velocemente al merito, il disegno di legge ha due principali obiettivi, il primo dei quali è riconoscere il valore del settore. L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli un patrimonio culturale da valorizzare e tutelare, con un'attenzione particolare alla qualità, alla certificazione geografica e di origine, ai vigneti cosiddetti eroici e storici, ai vitigni autoctoni, alle produzioni di nicchia, ai vari prodotti legati al vino ed al mosto cotto, ai succhi d'uva, all'aceto. Allo stesso tempo risponde al ruolo economico del settore, che costituisce la maggiore voce dell'*export* agroalimentare del Paese e uno dei simboli più importanti e caratteristici del *made in Italy*. Infine, il provvedimento intende mettere ordine in un panorama normativo molto complesso, condizionato da normative europee, nazionali, locali e regionali che hanno reso improcrastinabile una disciplina organica in grado di coordinarle ed armonizzarle, secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli anche in funzione di un'esigenza generale di certezza del diritto. Da qui l'introduzione dello schedario viticolo, le norme sulle certificazioni e il conferimento della protezione europea sulle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sui disciplinari di produzione, sui consorzi di tutela, sui concorsi enologici. Avendo deciso di non presentare emendamenti, se non quelli tecnici presentati in Assemblea, per favorire la rapida approvazione del provvedimento, la 9a Commissione ha recepito molte istanze presentate dai diversi Gruppi ed accolte anche dal Governo.

che oggi rinunciano a svolgere riflessioni e ad apportare ulteriori modifiche, dando invece priorità all'importanza del provvedimento e alle attese di migliaia di aziende del settore. Lo trovo un atteggiamento di grande responsabilità e maturità politica che fa onore a quest'Assemblea. Anche io consegnerò la parte della mia relazione che riguarda l'articolato e mi limiterò a sottolineare alcune novità di questo testo. La prima è il modo in cui il disegno da una proposta nata dentro la rappresentanza del mondo agricolo e imprenditoriale del vitivinicolo, che ha dimostrato come sia possibile svolgere un ruolo importante di proposta e non solo di singole rivendicazioni

ha aggiornato, semplificato, introdotto sistemi innovativi indispensabili nel tempo dell'informatica e della digitalizzazione. I punti cardine di questo provvedimento sono, appunto, la semplificazione delle procedure: semplificazione a partire dai sistemi di controllo. È questa la grande sfida del settore vitivinicolo e dell'agroalimentare in generale, non facile, significa essere capaci di semplificare le modalità e le procedure tenendo alto il rigore dei controlli; perché è sulla sicurezza, sulle garanzie di sicurezza alimentare che si basa la la reputazione del nostro sistema vitivinicolo, quindi strategia competitiva. Più efficacia dei controlli e meno complicazione significa raccordo tra gli organismi preposti ai controlli; significa banche dati del Sistema informatico nazionale (SIAN) che costruiscono, dato dopo dato, il profilo preciso, dettagliato, di ogni azienda; significa che potranno essere possibili interventi mirati, controlli anche a distanza, con minori viaggi, minori tempi, minori costi; significa riduzione di registri cartacei, riduzione di comunicazioni solo formali, cioè di quelle carte che certificano altre carte senza incidere sul processo reale. Una semplificazione che introduce finalmente il criterio di proporzionalità, come diceva il collega Panizza: non può esserci identico percorso di procedure, la stessa complessità per la grande azienda e la piccola impresa. Vengono introdotte norme specifiche in proporzione alla dimensione di produzione. Secondo grande principio che caratterizza tutto il provvedimento è la distintività come fattore competitivo e trasparenza insieme; quindi, un'informazione chiara degli elementi di distintività: una distintività misurabile, non solo basata su suggestioni. qui la definizione precisa di vitigno autoctono, l'indicazione precisa in etichetta della presenza di vitigni pregiati, se presenti in una percentuale fissata, limiti precisi alle dizioni di pregio classico, storico, riserva; più sistemi di trasparenza per la prima volta insieme al contrassegno di Stato per i vini di maggior pregio; vengono inseriti sistemi telematici di controllo anche ai vini di indicazione geografica, quelli di consumo quotidiano e di più grande diffusione commerciale, ma che puntano sempre più a qualità e sicurezza: uno strumento per i consumatori di maggiore conoscenza e informazione reale. Diversi i punti che riguardano strumenti e procedure che aumentano la tracciabilità del prodotto, informazioni sull'imbottigliatore quando non è indicato in modo preciso, l'obbligo di pubblicazione dei dati delle dogane sulle importazioni di vino, sulle imprese importatrici e le quantità, informazioni pubbliche. E dentro questo obiettivo, che tiene insieme qualità alta e maggiore semplificazione, si cerca di introdurre una logica nuova, cioè l'idea che sistema pubblico, mondo imprenditoriale e consumatori consapevoli possono essere alleati preziosi nella tutela della qualità, perché sicurezza e distintività sono fattori fondamentali per i insieme fattori competitivi strategici; l'idea che l'impresa non è il nemico di cui diffidare sempre e comunque, ma un alleato importante; l'idea che aumento di controlli non significa solo e sempre dispiegare più uomini ed eserciti, ma far maturare un controllo sociale, diffuso, di imprenditori che per primi difendono

ma anche un alleggerimento delle sanzioni e la possibilità di rimediare a errori solo formali, di carattere amministrativo, attraverso l'inserimento per la prima volta dell'istituto del ravvedimento operoso: la possibilità di regolarizzare pagando solo un ottavo delle sanzioni previste. Naturalmente è impossibile elencare qui tutte le misure del provvedimento, che sono anche molto tecniche, ma credo sia più importante per quest'Assemblea cercare di cogliere il senso complessivo del provvedimento, gli elementi di novità, lo spirito che accompagna questo testo; dare la consapevolezza a tutti noi dell'importanza economica che ha assunto il settore vitivinicolo nel nostro Paese. Un *export* che ha superato i cinque miliardi di euro, un fatturato di oltre 12 miliardi complessivi, che con l'indotto, raggiunge i 20 miliardi. Il nostro è il primo Paese produttore al mondo di vino, con imprese agricole di trasformazione, industrie, che coinvolge un tessuto sociale di oltre cinque milioni di persone. È un comparto che rappresenta un settore economico con prospettive di nuova occupazione, di nuove professioni; è un pezzo grande del nostro futuro, ma credo che lo possa essere se non suddividiamo numeri e fatturati dagli altri tratti del settore del vino, che sono territorio, cultura, salute e sapere insieme. Per questo credo che il cuore del provvedimento stia, in modo non retorico, proprio nel Capo

di assecondare questo provvedimento in quanto lo stesso è stato sostanzialmente costruito assieme al settore vitivinicolo. Purtroppo da tanti anni si attendeva un provvedimento che fosse capace di inquadrare nel suo insieme tutte le normative legate alla produzione vitivinicola, dalla tutela dei marchi fino alle norme e alle garanzie di produzione. Questo provvedimento ha in sé molti, se non tutti gli elementi che occorrono per dare soddisfazione a queste richieste. Signor Presidente, è importante anche fare una sottolineatura, vista la situazione politica e anche il prossimo *referendum* del 4 dicembre. infatti, ci troviamo nella curiosa condizione di modificare il testo in quanto nello stesso è contenuto un errore che è sfuggito all'approvazione della Camera dei deputati.

con una consapevolezza: nulla c'entra il bicameralismo con la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle leggi. Semplice: se le leggi vengono scritte bene, che siano approvate da una o due Camere nulla cambia; se le leggi sono scritte male, come in questo caso, purtroppo con un errore, la seconda lettura consente e sta consentendo di poter modificare, impedendo che addirittura possano esservi pregiudizi per alcuni produttori riguardo all'emanazione di un provvedimento di legge. Non entro nei termini del provvedimento stesso, signor Presidente, proprio perché non voglio dilungarmi. Noi abbiamo auspicato la tutela e la difesa della qualità del *made in Italy*.

molto in termini di quantità riescono a fatturare moltissimo di più, quasi un terzo in più se non il doppio in alcuni settori, in termini di valore del prodotto nella quantità unitaria. quindi, spingere il nostro settore non solo alla quantità prodotta, ma anche alla qualità e soprattutto alla promozione e alla consapevolezza del valore del vino*made in Italy*. Italy*. In alcuni Paesi - penso agli Stati Uniti - il vino francese è da sempre considerato molto più del vino italiano, purtroppo; questa è una carenza nella coscienza e nella diffusione del *made in Italy*. Bisogna impegnarsi molto di più, quindi. A partire da queste norme e da queste regole, l'impegno che il Governo deve prendere è di sostenere la promozione del prodotto nazionale più qualificante e certamente più apprezzato nel mondo.

G28.100, naturalmente associandomi alle considerazioni sulle positività di questo disegno di legge e sul fatto che è atteso in maniera particolarmente positiva da tutto il comparto. Il mio ordine del giorno tende a salvaguardare la specificità del consorzio di tutela del vino Marsala. Si tratta dell'unico consorzio di tutela

Purtroppo, alla lettura del decreto legislativo che regola i consorzi di tutela sembrerebbe che, non essendo il vino Marsala corrispondente ai cosiddetti vini di base ma essendo solo frutto di una lavorazione assolutamente rigorosa e specifica disciplinata

pertanto il Governo e l'Assemblea di considerare positivamente la necessità che anche il consorzio di tutela del vino Marsala possa rientrare tra i consorzi di tutela previsti dall'articolo 41 della normativa.

Mi limito a sottolineare l'importanza del provvedimento e la sua grande rilevanza per un settore che è davvero trainante per l'economia del nostro Paese.

fatto che, obiettivamente, andiamo a rendere onore a una grande filiera e a metterla nella condizione di poter, a brevissimo, avere una legge attesa da molti anni.

considerando il caso della denominazione di origine controllata Marsala, eventualmente anche stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base.

Presidente, più che consegnare il testo, farò una dichiarazione di voto asciutta e sobria. Signor Presidente, per noi il vino è tutela del territorio, per il mercato, è tutela dei marchi. Su questo esiste una differenza fondamentale e lo diciamo al Governo. L'impegno che il Governo deve assumere in attuazione di questo provvedimento è la promozione del nostro territorio, che significa promozione del vino.

Occorre, però, che alle normative (come alle Costituzioni) sia data poi attuazione. Al Governo lasciamo quindi questo impegno, su cui vigileremo in maniera molto serrata, perché il settore sia sostenuto, fiscalmente ed economicamente, con una promozione che consenta ai nostri produttori quella competitività che già di per sé la qualità del vino meriterebbe, ma che merita ancora di più in ragione dell'impegno che mette tutta la filiera nella produzione delle eccellenze vitivinicole italiane. Signor Presidente, sarò davvero brevissimo. Non ho documenti da consegnare, ma vorrei fare una dichiarazione molto succinta

della brevità del mio intervento: la prima è la sburocratizzazione e, quindi, la semplificazione di alcuni adempimenti che, nel tempo, erano diventati un ostacolo

due principali ragioni per le quali il mio Gruppo voterà convintamente a favore di questo provvedimento. L'ultima nota riguarda l'ordine del giorno G28.100 presentato dal senatore D'Alì

i produttori (ma non solo) chiedevano l'approvazione di questo riordino e di questa disciplina organica, peraltro importante sia dal punto di vista

anche io aderisco volentieri al suo invito e quindi consegnerò il testo del mio intervento, ma ho il dovere di esprimere in Aula l'adesione convinta di tutto il Gruppo a questo testo unico

accendere un faro sul dato diffuso da Coldiretti: l'Italia è il primo produttore mondiale di vino, con in media 47,5 milioni di ettolitri ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati. Il vino, perciò, si eleva a prodotto agroalimentare italiano più esportato: un volume di affari di 5,4 miliardi di euro, dove l'Italia spicca a livello europeo per varietà di uva da vino (453 nel totale), e per vini a denominazione di origine, 73 sono DOCG, 332 sono DOC e 118 sono IGT. Parliamo di un'industria che non solo conta su una cospicua varietà di vitigni, ma che rappresenta - a livello internazionale - uno dei tratti maggiormente caratterizzanti del nostro Paese, perché coniuga il buono (quello delle eccellenze enogastronomiche) con il bello (quello dei nostri paesaggi rurali e della connessa eredità culturale e storica). Non è un caso che proprio l'Italia sia destinazione privilegiata di tantissimi estimatori, studiosi, imprenditori, ma anche luogo di antiche pratiche enologiche. Spiegate le premesse di uno dei fiori all'occhiello del comparto agricolo ed enogastronomico nazionale, questo provvedimento si propone di razionalizzare le numerose disposizioni interne riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Un testo che gli operatori del settore aspettavano da tempo e che - speriamo - li sollevi una volta per tutte da inutili oneri burocratici e norme criptiche, nemiche della semplificazione, quella che dovrebbe evitare di perdersi tra rimandi senza capo né coda. Sì, perché il vino, la vite e i territori viticoli non sono semplicemente una componente di un comparto; sono anche e soprattutto parte del nostro patrimonio che, come tale, deve essere valorizzato nelle sue diverse declinazioni. La valorizzazione della filiera del vino, però, implica, prima di tutto, la sua protezione. Ci sono svariati elementi che influiscono negativamente nella coltivazione e successiva produzione. Non solo fattori climatici ed ambientali come piogge, gelate, grandini, ma anche agenti patogeni. A tal proposito, a settembre di quest'anno, la Puglia è stata interessata, insieme ad altre Regioni, da un *mix* letale: condizioni climatiche avverse accompagnate dalla pericolosa diffusione della botrite, la cosiddetta muffa grigia della vite. Sul punto, lo scorso 3 ottobre, numerose amministrazioni locali pugliesi, del barese e del foggiano - da Noicattaro a Bitetto a Rutigliano hanno inviato una espressa richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione Puglia e agli organi di Governo. insieme alle alte temperature tipiche del periodo, hanno fatto sì che si creassero le condizioni per lo sviluppo di patologie fungine a scapito di molti prodotti agricoli. Si è dovuto perciò procedere alla rimozione degli acini colpiti dalle malattie fungine, con un aggravio delle spese per i territori. In altri casi è stata necessaria la raccolta dell'intera produzione da destinare all'estrazione di succhi o di saccarosio, con un prevedibile crollo del prezzo di vendita del prodotto a centesimi di euro. Ma non solo la Puglia è stata vittima di questi eventi; anche altre Regioni d'Italia. Ricordo, ad esempio, i danni ai vigneti del Chianti classico, Montalcino e Montepulciano, di cui si è molto parlato nei mesi scorsi.

Vale la pena sottolineare, poi, che non solo la botrite affligge le piante di vite. C'è il cosiddetto mal bianco, che si manifesta con macchie feltrose bianche su foglie e con gli acini che si spaccano o fessurano.

Detto questo, nonostante il provvedimento ci trovi sostanzialmente favorevoli, abbiamo voluto precisare alcuni aspetti. Vale la pena rimarcare che su questi punti il Governo si è già impegnato, perché si tratta di nostri ordini del giorno approvati in Commissione agricoltura. Parliamo di percorsi che stiamo portando avanti passo dopo passo e che segnano la nostra idea di agricoltura con delle precise parole chiave: sostenibilità, biodiversità, tutela del *made in Italy* e della filiera corta, tracciabilità. Partendo quindi dall'ambito regionale, il Governo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, dovrà adottare ogni provvedimento utile a sostenere e incentivare le imprese pugliesi che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie. Ricordiamo che la Puglia è una Regione da sempre ai vertici nel campo e di certo non può rimanere vittima dei cambiamenti climatici. Ricordo il caso della frode della Per questo, non bisogna mai dimenticare che i sostegni vanno indirizzati proprio in questa direzione. E per questo ci siamo battuti affinché si desse particolare attenzione al Primitivo di Manduria, un vino DOC conosciuto in tutto il mondo, la cui produzione è consentita nelle Province di Brindisi e Taranto. Abbiamo chiesto di tutelare, partendo da una difesa ambientale, quei territori che producono questo vino, ma anche le aziende che operano nell'area. A livello nazionale, poi, abbiamo richiesto e ottenuto un chiaro impegno volto alla promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sui prodotti vitivinicoli, al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su prodotti di qualità. È necessario, poi, favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Ogni giorno arrivano sulle nostre tavole tantissimi prodotti di cui non conosciamo la provenienza e che spesso celano malaffare, frodi agroalimentari, storie di sfruttamento. Per questa ragione, da sempre, chiediamo un macro-sistema di tracciabilità degli alimenti affinché ogni consumatore possa conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di ciò che mangiamo, che beviamo, che troviamo negli scaffali del supermercato. Sul punto, nello specifico, c'è una proposta a mia prima firma che reca norme per la tracciabilità dei prodotti agricoli. Ancora, nelle opportune sedi, l'Esecutivo dovrà promuovere - in tutte le sue forme - la salvaguardia del vero *made in Italy* anche in tema di vini, se necessario - del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa riguardante le etichettature. Questa mattina abbiamo visto la presentazione di tre emendamenti volti in questo senso. Per fortuna - ribadiamo ancora una volta - che esiste il Senato della Repubblica! Il Senato, che ha accolto il suggerimento da parte della Commissione giustizia e che ha potuto, quindi, sistemare la normativa e portare un buon risultato. Quindi io dico "no" alla riforma costituzionale anche per questo motivo. È ora che il tempo impiegato in farraginose procedure burocratiche, adempimenti spezzettati e passaggi disorganici lasci il passo alla dematerializzazione, alla riduzione dei tempi e dei costi, in un contesto in cui non esiste più una quantità indefinita di discipline, ma ce ne è una sola ed è quella del testo unico sul vino. Parafrasando una frase di Galileo Galilei,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi debbo dire che abbiamo assistito a una volontà praticamente unanime nell'esprimere, attraverso un voto altrettanto

il nuovo continente, gli Stati Uniti.

Noi ci siamo, i viniviticoltori ci sono. Non ci sono altri come lo siamo noi. C'è molto lavoro da fare in questo senso.

Il settore procede e cresce non senza difficoltà, perché dire che tutto va bene sarebbe sbagliato. Abbiamo - mi ripeto volutamente - una grande responsabilità, quella di essere presenti nel mondo con un prodotto di eccellenza e aspirare a esserlo sempre di più, con un *brand* che ci caratterizza, ossia il vino *made in Italy*. Attenzione, i pericoli

della semplificazione e della sburocratizzazione, dovrebbe essere seguito anche in altri settori. L'unanimità cui siamo arrivati è proprio il frutto della

che il settore ha fatto con fatica, serietà e dedizione negli ultimi anni e che lo ha portato a essere *leader* nel mondo.

«per quanto sopra premesso e considerato impegna il Governo a valutare la possibilità che, in occasione di una disciplina organica della materia, si adottino misure volte a garantire l'informazione al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da rispettarne l'autonomia e la dignità».

al comma 3 specifica che «Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con poteri e modalità stabilite dalla legislazione regionale».

sull'emendamento 2.203, che peraltro, come giustamente richiamato, giustifica il parere contrario dato

dell'articolo 3, aggiunge le parole: «e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure», laddove si individuano le misure che devono essere assunte con riferimento ai riferimento ai dati raccolti nell'ambito del percorso di formazione tra strutture sanitarie, centro regionale e osservatorio. Sostanzialmente l'Osservatorio acquisisce una funzione che attiene non solo alle linee di indirizzo individuate in base all'adozione delle misure di prevenzione per la gestione del rischio, ma anche alle linee finalizzate al monitoraggio delle buone pratiche

sulla sicurezza nella sanità», in conseguenza dell'emendamento che è stato approvato e che evidentemente non ha indotto

che, qualora un medico disponga l'autopsia, ai familiari sia consentito che un loro medico di fiducia possa partecipare

Perché non gli è consentito? Perché la legge non lo prevede, per un quadro peraltro piuttosto complesso, per una visione piuttosto pubblicistica del cadavere e non per una visione privatistica. L'unico modo per far sì che un familiare abbia un suo medico presente all'autopsia è di fare una denuncia. Nella mia esperienza di un piccolo ospedale mantovano, in pochi anni, acconsentendo che i familiari potessero mandare un loro medico di fiducia, ho evitato una decina di denunce. Oggi voglio ricordare che un pubblico ministero, quando si trova di fronte a cartelle impegnative, non fa altro che prendere i nomi di tutto il personale e inviare loro un avviso di garanzia.

Un familiare può andare da un professionista, pagare anche 800-1.000 euro per una visita, ma non può chiedere un'autopsia, che ha un costo di 380 euro, perché tanto è valutata l'autopsia anche in ambito giudiziario per un perito.

- dopo il comma 3, con riferimento all'accesso alle informazioni relative alla documentazione sanitaria in possesso

in relazione alla necessità che l'obbligo di trasparenza consenta sia al medico che alla struttura sanitaria di poter provare il cosiddetto corretto adempimento tramite la documentazione sanitaria relativa alle prestazioni effettuate anche al di fuori della struttura utilizzata dal paziente.

al trattamento sanitario che il danneggiato ha avuto relativamente alla patologia per la quale si è determinata la richiesta di risarcimento. Questo è il motivo per il quale chiedo un'attenzione supplementare da parte del Governo e del relatore. Credo che questo emendamento sia perfettamente in linea con i principi della trasparenza che non possono essere sbilanciati, ma devono mantenersi in una condizione di equilibrio. **Saluto finestra"). Onorevoli colleghi, salutiamo il sindaco e la delegazione della Giunta del Comune di San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori.

«impegna il Governo a valutare le modalità - è questo il problema - per introdurre la possibilità per i familiari (o gli aventi titolo) di

invece un parere favorevole sull'ordine del giorno che è impegnativo per il Governo.

e, anche sui siti delle *big pharma*, i soldi che hanno percepito. È molto interessante notare come, all'estero, questi eminenti colleghi dichiarino conflitti di interesse, mentre in Italia non lo facciano.

Voglio ricordare che all'estero questo è un problema molto importante, e ciò è tanto vero che gli inglesi hanno costituito l'istituto NICE, che riceve finanziamenti pubblici per 33 milioni di sterline all'anno

sul «British Medical Journal del 2016», nell'ambito dei quali si dimostra che più le società scientifiche sono grandi, più hanno grande potere, più hanno grandissime sponsorizzazioni.

Il relatore ha posto una serie di elementi che, tutto sommato, non godono della mia completa fiducia, ma riconosco il suo lavoro e, senza fondi, più di questo non si poteva fare.

dell'elaborazione delle linee guida, introduce un tema importante, vale a dire quello delle federazioni e gli ordini. Vorrei fare una riflessione al riguardo e un passo indietro. Abbiamo tutti votato il disegno di legge del ministro Lorenzin che ribadisce agli ordini un ruolo di enti di diritto pubblico. Credo davvero sia importante che, nell'elaborazione delle linee guida, debba essere assicurata la partecipazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici, della Federazione nazionale collegi infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e delle altre federazioni nazionali collegi delle professioni sanitarie. Se qualche settimana fa abbiamo riconosciuto

ai singoli cittadini e ai singoli comitati. Diamo a Cesare quel che è di Cesare: non ci si laurea, non ci si specializza, non si fanno venti, trenta, quarant'anni di studi nelle università - validati con metodo e linee guida anche nella metodologia di scrivere un lavoro e di portarlo avanti -

(si spera meritocratica), una specializzazione altrettanto meritocratica e abbia effettuato un percorso personale di studio, di aggiornamento ed esperienze, che che pure hanno un peso. Quindi, diciamo che le linee guida servono, alla luce dei metodi validati, dei *gold standard* e delle ultime ricerche,

dal momento che non è stato specificato bene nel provvedimento quali sono le società scientifiche, gli enti, le istituzioni pubbliche o private, vorrei capire se le federazioni presentato dal collega Mandelli, il 5.210, si intendono già comprese nelle società da consultare per l'emanazione delle linee guida o se ne sono escluse.

prevede che il Ministero ridefinisca nella composizione e nelle funzioni il sistema nazionale delle linee le modalità con cui questo organismo provvederà a interloquire con tutte le competenti autorità scientifiche e professionali.

tutte quelle partecipazioni, comprese quelle dei gruppi multidisciplinari di cui si parlava prima. È questa la *ratio*. È una norma primaria, che dà indirizzi

tener conto dei gruppi multidisciplinari. Si farà in modo che si tenga conto di tutto questo. la legge n. 42 del 1999 già prevedeva, nell'allora sistema nazionale linee guida, la partecipazione di federazioni degli ordini.

confermo che sarebbe molto complicato dettagliare tutti gli spunti che vengono qui indicati in una norma primaria.

non economici e il loro *status* giuridico è reiterato dall'articolo 3 del cosiddetto disegno di legge Lorenzin, all'esame della Camera

È scritto espressamente che le linee guida sono elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati. poiché gli ordini hanno una natura giuridica che li qualifica come enti di diritto pubblico, sono

stabilite dal decreto del Ministero cui l'articolo 5 fa riferimento. Mi sono permesso di fare questa precisione, perché la puntualizzazione nel Resoconto potrà dirimere qualche dubbio ed eliminare incertezze nell'ambito dell'interpretazione.

ovviamente - non entrano nel merito. Siccome noi facciamo dipendere la non punibilità anche per errore grave dall'aver seguito le linee guida, chiedo al relatore

dal punto di vista tecnico-scientifico (ma devo dire prontamente anche sotto quello giuridico), che le linee guida sono delle raccomandazioni

e adeguate al caso concreto. Questo lo ha già detto anche la magistratura: ci sono sentenze che condannano professionisti per un rispetto acritico - come dice la magistratura - delle linee guida. È una materia molto complessa. L'importante però